la seguente lettera: «Roma, 7 novembre 2016, Illustre Presidente, Le comunico che in data odierna la Corte, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento generale, ha accettato le dimissioni dell'avvocato Giuseppe FRIGO che, pertanto, in pari data cessa dall'ufficio di Giudice costituzionale. *F.to* Paolo Grossi». Onorevoli colleghi, nella serata di ieri è mancato Umberto Veronesi, oncologo e studioso di fama mondiale. Nato a Milano il 28 novembre 1925, dopo aver conseguito la laurea in medicina e chirurgia, si specializza nella ricerca e nella cura delle patologie tumorali: inizia così la sua collaborazione, come volontario, presso l'Istituto nazionale dei tumori, di cui di diviene direttore generale nel 1975. Contribuisce alla fondazione dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro e della Scuola europea di oncologia; dal 1985 al 1988 presiede inoltre l'Organizzazione europea per la ricerca e la cura del cancro. Fonda inoltre l'Istituto europeo di oncologia. È stato Ministro della sanità nel II Governo Amato. Viene eletto al Senato nel 2008. Nel febbraio 2011 si dimette da senatore, per ricoprire l'incarico di presidente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare. Il suo contributo intellettuale

propria di un uomo che ha contribuito alla cura e alla salvezza di tantissimi pazienti. Il suo lascito intellettuale è rappresentato dall'ultimo messaggio reso noto ieri dalla Fondazione omonima: «Andate avanti, perché il mondo ha bisogno di scienza e ragione». Raccogliendo idealmente questa esortazione dell'uomo, prima ancora che dello scienziato, il Senato della Repubblica si unisce al dolore della famiglia e della comunità scientifica. Invito quindi l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri i relatori hanno illustrato i documenti. Dichiaro aperta la discussione congiunta. È iscritta a parlare la senatrice Padua. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento riguarderà soprattutto la parte della relazione che interessa la Sicilia e d'altra parte, permettetemi, non potrebbe essere altrimenti. La portata della crisi che riguarda la Sicilia nel settore dei rifiuti emerge in modo lampante dall'attività e dalla relazione della Commissione di inchiesta. Nel documento, infatti, si parla diffusamente di sistema di

infatti, si parla diffusamente di sistema di illegalità diffuso e radicato che costituisce uno dei veri ostacoli per la risoluzione delle problematiche esistenti,

di strumenti per combattere le emergenze che si sono rivelati inefficaci e controproducenti: sono parole drammatiche e dolorosissime; sono pietre e sono scritte nella relazione. Il quadro complessivo che emerge dai lavori e dagli accertamenti compiuti sul sistema della gestione dei rifiuti siciliano è, a dir poco, estremamente preoccupante, sia per l'emersione e la presa d'atto dell'incapacità della Regione, nel presente e nel passato, di far fronte e gestire le emergenze, sia (fatto ancor più grave) per la palese dimostrazione di incapacità nella programmazione e nel governo dei processi e delle scelte per un rinnovamento. La Commissione ci ricorda come a partire dalla prima dichiarazione dello stato di emergenza, stabilita in un'ordinanza dal Presidente del Consiglio dei ministri nel 1999 per superare l'esistenza di una discarica in ogni singolo Comune e introdurre un sistema di gestione conforme con la normativa nazionale anche in materia di raccolta differenziata, la situazione non sia affatto migliorata. D'altra parte mi chiedo perché dovrebbe crescere la raccolta differenziata se i responsabili sono gli stessi che gestiscono le discariche? Quale motivazione potrebbe mai spingerli ad abdicare ai propri interessi? Anzi, al contrario, a partire dal 2002, l'idea di costruire mega inceneritori non ha fatto altro che compromettere lo sviluppo della raccolta differenziata, rimasta ferma, e la costituzione degli ambienti territoriali ottimali ha escluso i Comuni dalle scelte sulla gestione, lasciando governare il tutto a società e persone che hanno tratto benefici, a discapito delle comunità locali, da una sequenza di processi oscuri, concatenati tra loro. Ne sono rimasti investiti profili che riguardano la sicurezza e la salubrità delle persone e dei territori, con discariche spesso non messe in sicurezza e con la presenza di percolato che certamente ha determinato gravissimi danni alla vegetazione e agli animali e, potenzialmente, alla salute delle persone. Processi di mala gestione che sono partiti e si sono sorretti sui mancati controlli da parte della Regione e sulle modalità distorte con cui sono state rilasciate le autorizzazioni per le discariche private. Tramite tale *modus operandi* si è alimentato lo sviluppo di percorsi illeciti e malavitosi. Il fatto che si possa «ragionevolmente presumere una permanente deviazione delle funzioni pubbliche in favore di imprese private operanti nel settore dei rifiuti», come viene detto nella relazione, perché gli uffici occupati al rilascio delle autorizzazioni si sono dimostrati corrotti oltre ai recenti tentativi messi in atto per riformare l'assetto delle competenze sulle procedure per la valutazione e il rilascio dell'AIA stanno a palesare chiaramente il fallimento complessivo di un sistema che in luogo della buona fede, della trasparenza e del possesso di adeguate conoscenze, ha strutturato l'azione congiunta degli apparati politico-amministrativi sull'interesse di parte. Il Governo in carica, purtroppo, non è riuscito a dare la necessaria sferzata a tutto questo, tanto che attualmente, si legge nella relazione: «molti territori siciliani sono invasi dal pattume e l'idea di portare i rifiuti fuori regione è la prova più lampante dell'attuale crisi di sistema». Eppure, nel grigiore e nella bassezza della rappresentazione di un quadro che è un crescendo di desolazione, la speranza e la prospettiva di una svolta positiva non possono spegnersi. La speranza è quella che i processi sulla gestione dei rifiuti siano affidati alla cura di persone serie e competenti, che pongano a fondamento delle proprie scelte il bene di questa meravigliosa isola che è la Sicilia e quello delle future generazioni. È verso di loro, in primo luogo, e verso la custodia di un bene, l'ambiente, che è patrimonio comune, che bisogna esigere, come classe politica, un cambio di direzione, di mentalità. Il rinnovamento deve riguardare *in primis* la cultura della classe politica, amministrativa e professionale locale ma, per riuscire, deve saper coinvolgere tutte le componenti del sistema:

Se un'emergenza è cronica, chiaramente, non può più essere definita tale e in Sicilia passiamo da un'emergenza all'altra senza riuscire mai ad uscirne. Dunque il problema è strutturale e come tale va affrontato. Della funzione supplente della magistratura nei riguardi dell'amministrazione regionale per ricondurre il sistema della gestione dei rifiuti nei confini della legalità va dato atto. Tuttavia, senza un impegno politico complessivo e certo non si riuscirà a fare quel primo passo che è imprescindibile per delineare un vero cambiamento: una programmazione ordinaria e realistica che bilanci le esigenze di non far collassare il sistema e di strutturare percorsi idonei a risolvere una questione incancrenita, ritrovando nell'ordinarietà e nel rispetto della legalità il migliore viatico d'uscita.

Siciliana, partendo dal Veneto. Il documento proposto dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti riguardante la situazione territoriale della Regione Veneto, è frutto di un lavoro interessante, delicato e sicuramente meritevole di analisi. Così come è ben descritto anche nella approfondita relazione presentata, la regione Veneto si contraddistingue per diversi aspetti, addirittura paradossali o meglio contraddittori, primo tra tutti la convivenza in un territorio circoscritto di ben 1.500 impianti per il trattamento di rifiuti speciali, molte volte oggetto di indagini giudiziarie, con una realtà lodevole in materia di smaltimento di rifiuti perché tra le più virtuose d'Italia. Le vicende giudiziarie hanno riguardato alcuni dei più rilevanti scandali ambientali veneti: dai rifiuti di Marghera, impastati sotto la rampa dell'autostrada di Roncade a Treviso, alle scorie di acciaieria smaltite sotto al parcheggio P5 dell'aeroporto Marco Polo di Venezia, fino alla forestazione della discarica di Sant'Urbano a Padova. Una prima amara valutazione che viene fuori, quindi, è che anche il Nord-Est - e non solo il Sud

di Venezia, trova radicamento in un atteggiamento di diffusa omertà tra gli operatori economici. Non è un caso come nella Regione Veneto si contino 485 siti contaminati tra i quali vanno ricompresi numerosi siti nei quali, per lunghi anni, le società hanno gestito illecitamente rifiuti speciali anche pericolosi e che, dopo il sequestro degli impianti da parte dell'autorità giudiziaria, sono state dichiarate fallite lasciando a carico degli enti territoriali i costi, anche per molte decine di milioni di euro, connessi alle attività di allontanamento dei rifiuti pericolosi, di messa in sicurezza

vi è la pratica del cosiddetto giro bolla, cioè dell'operazione di sostituzione del documento originale di accompagnamento di un rifiuto contenente un determinato codice CER, con uno riportante indicazioni false. Una particolare menzione merita inoltre la vicenda dell'inquinamento delle acque da PFAS, sostanze perfluoroalchiliche, provenienti dalla azienda Miteni di Trissino in provincia di Vicenza. Un grave inquinamento da sostanze persistenti, i PFAS, che oramai sono entrati nel ciclo alimentare, interferendo negativamente sul metabolismo animale e umano. La diffusione di queste sostanze va quindi prevenuta in tutti i modi possibili. Passo ora a qualche commento sulla relazione riguardante la Regione Siciliana. Il documento proposto dalla Commissione parlamentare d'inchiesta relativo alla Regione Siciliana è decisamente più problematico. L'incredulità nel leggere quanto emerso da questa relazione trova giustificazione non solo perché viene chiaramente denunciata e certificata l'emergenza per la gestione dei rifiuti, ma perché è avvalorata dalla commistione esistente tra smaltimento rifiuti e criminalità organizzata. Da parlamentare fa tristezza leggere una chiara responsabilità dei funzionari pubblici nella gestione dello smaltimento di rifiuti, ancor di più se in presenza di incapacità amministrativa e fenomeni corruttivi. Sono pagine piene di casi di inerzia o di inadempienza, di corruttele e di sotterfugi amministrativi. Sono pagine che sanciscono il fallimento della politica come responsabile del bene pubblico e dell'inevitabile supplenza della magistratura per una gestione fallimentare nei confronti della propria morale e di qualsivoglia etica lavorativa. La situazione emergenziale che caratterizza la Regione Siciliana deve responsabilizzarci di fronte a quella che è stata una mancanza di volontà, politica e amministrativa. Già la gestione commissariale siciliana, cominciata nel lontano 1999, è stata una colossale macchina di denaro a vantaggio dei trasportatori e dei proprietari di discariche. Nondimeno, la fase emergenziale non ha mai prodotto una rete impiantistica e di smaltimento degna di questa situazione, gravando di fatto in termini di costo sul sistema ATO. Si sono costituiti 27 ATO, che hanno esautorato la responsabilità dei Comuni: un'operazione fallita, sia dal punto di vista economico che politico. A questo punto concordo in pieno con la decisione del Governo di non prolungare e non dare non dare un ulteriore commissariamento. È stato più saggio impartire delle direttive e delle indicazioni, anche se, ad oggi, non c'è ancora una vera programmazione. Ad esempio, nella relazione viene chiaramente denunciato come, su ben novantotto centri comunali di raccolta, realizzati alla data del 2010 grazie alle risorse provenienti dalla programmazione europea (POR 2000-2006), oltre il 50 per cento di questi o non era autorizzato o non era in attività. Come è possibile, mi chiedo? Sorgono preoccupanti dubbi relativamente alle modalità con le quali si è proceduto ai colludi e alla certificazione della spesa comunitaria, visto che, tra le condizioni necessarie a garantire l'ammissibilità del finanziamento, vi erano il progetto

non è opportuno, anche nel rispetto del lavoro svolto dalla Commissione d'inchiesta. La Sicilia vive una quotidiana situazione di emergenza sia con riferimento alla situazione delle discariche che a quella economica che ne è derivata. Signor Presidente, le mie riflessioni non potevano quindi che essere amare e cariche di rabbia. Una rabbia però - spero - positiva, perché non possiamo tacere di fronte a tanta inefficienza e incapacità. Quella che stiamo esaminando è una relazione sulla verità, una verità che per molto tempo non abbiamo affrontato con il giusto rigore. Diamo, però, un messaggio positivo cittadini siciliani, affinché le nostre valutazioni non rimangano anch'esse solo sulla carta.

ciò che riguarda i rifiuti: autorizzare un percorso di smaltimento che sia di interesse nazionale, perché la crisi di tutte le Regioni sui rifiuti molto spesso si traduce in un aumento dei e dei costi, soprattutto per le successive bonifiche. Bisogna interrogarsi su come intervenire effettivamente per semplificare e coordinare. Questo è il percorso che l'Italia deve affrontare, insieme alle idee e alle pratiche di economia circolare, ma anche sulla base di concetti di riduzione della produzione del rifiuto. Si tratta di un percorso a medio termine importante, virtuoso e da portare avanti necessariamente. Tuttavia, nella drammaticità della problematica immediata che coinvolge tutte le Regioni, l'intervento a livello nazionale di coordinamento e di gestione integrata del problema dei rifiuti deve essere un percorso da portare avanti con caparbietà. Se l'obiettivo principale del Governo e del Parlamento deve essere rappresentato dalla tutela dell'ambiente e dalla salute di tutti i cittadini, penso che le relazioni in esame siano l'occasione per farci aprire gli occhi e che il nostro voto possa essere uno stimolo a risolvere le questioni evidenziate dalla Commissione. In conclusione, ringrazio i relatori, i collaboratori e i consulenti della Commissione per le relazioni, che ritengo esaustive e ben fatte, - non di meno - mettono in luce con coraggio quanta difficoltà ci sia nella gestione dei rifiuti e, purtroppo, anche la connivenza con il malaffare. *(Applausi colleghi, come sottolinea la Relazione, il SIN di Bussi sul Tirino rappresenta un esempio di quello che la Commissione sta evidenziando nelle sue inchieste, cioè di un insediamento in cui, nel corso di molti decenni, si sono svolte attività industriali pesanti nel settore della chimica che, venute progressivamente a cessare, hanno lasciato un sito contaminato. Se la relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti impegna il Governo, per quanto di competenza, ad intraprendere ogni iniziativa utile al fine di risolvere le questioni evidenziate nella relazione, le stesse iniziative non possono dimenticare, proprio per essere efficaci nelle risposte, le responsabilità. Bussi è uno dei quaranta siti nazionali per le bonifiche, cioè una delle aree più inquinate d'Italia e d'Europa, sede di un polo chimico dal 1902 dove, negli anni Trenta del secolo scorso, si producevano anche armi chimiche. Per circa vent'anni 700.000 cittadini della Val Pescara hanno bevuto acqua contaminata e solo la denuncia delle associazioni presentata nel 2007 ha fatto chiudere questi pozzi. Proprio nel 2007 è stata scoperta la cosiddetta megadiscarica dei veleni: una superficie di circa 30 ettari dove sono state intombate quasi 250.000 tonnellate di rifiuti tossici e scarti industriali, una bomba ecologica al confine tra il Parco del Gran Sasso e quello della Maiella, proprio a Bussi sul Tirino, in Abruzzo. Una vicenda che ha visto, in una discussa sentenza, assolti per prescrizione nel 2014 19 persone, tra ex amministratori, ex dirigenti e tecnici dell'azienda chiamati a rispondere di disastro ambientale. Su Bussi la parola «disastro» riguarda non solo quanto accaduto all'ambiente, ma anche lo stato delle istituzioni del Paese: questo è quanto dichiara il Forum abruzzese dei movimenti per l'acqua, che ha divulgato la relazione che conferma la fuoriuscita di decine di sostanze tossiche e cancerogene da tutte le aree del sito, dall'area industriale alla discarica Tremonti. Non possiamo dimenticare il pesantissimo impatto sull'ambiente e sulla salute che continua ad avere il sito della ex Montedison. Come ha denunciato il Forum illustrando i contenuti di uno studio ufficiale dell'Istituto zooprofilattico Abruzzo e Molise sull'ecosistema del fiume Aterno-Pescara, la pesantezza dell'impatto sta nel fatto che le sostanze tossiche rilasciate per anni dal sito di Bussi sono purtroppo entrate nella catena alimentare. Il mercurio supera i limiti di legge in un pesce su tre tra quelli pescati a valle del sito di Bussi sul Tirino, in provincia di Pescara, dove l'esposizione a sostanze tossiche è cronica, poiché la presenza dei micronuclei non si manifesta più dopo la depurazione e, quindi, potrebbe derivare da falda inquinata o da scarichi non trattati ancora attivi con continuità. Come è stato ricordato a suo tempo dal Forum per l'acqua Abruzzo, Bussi rappresenta ed ha rappresentato allo stesso tempo un disastro informativo, perché sono stati i cittadini a far uscire i documenti e ad informare la cittadinanza, quando invece il decreto n. 195 del 2005 impone da ben undici anni agli enti di pubblicare *online* i dati dei monitoraggi ambientali. È stato inoltre un disastro tecnico, amministrativo e giudiziario, un prototipo di disastro. Insomma, sono mancati il raccordo e la leale collaborazione tra i competenti organismi nazionali, le Regioni e gli enti territoriali interessati, che ci consegnano questo disastro. È tempo ormai di curare le cause e non solo i sintomi. In tal senso, noi daremo forza con il nostro voto alla risoluzione congiunta. L'auspicio è che il Parlamento, chiamato a trattare sulla salute dei propri concittadini, stavolta si senta libero. Noi tutti, espressione della popolazione, dobbiamo lavorare per ripristinare la normalità e far vivere in sicurezza i cittadini, che hanno pagato e continuano a pagare pesantemente Governi scellerati come questo, sottomessi alle multinazionali di turno. PRESIDENTE.

la relazione territoriale sulla Regione Veneto e la relazione territoriale sulla Regione Siciliana. Per quanto riguarda il Veneto, viene fuori una fotografia interessante, perché sicuramente si tratta di una Regione che da decenni ha saputo curare con grande attenzione il settore, disegnando quindi una sorta di eccellenza dal punto di vista territoriale, con un sistema di raccolta secco-umido che interessa il 99 per cento Ma quello che viene fuori - ed è molto interessante - è che la potenzialità complessiva degli impianti esistenti in Veneto è quasi doppia rispetto al fabbisogno regionale del trattamento dell'organico. Pertanto in questa Regione è venuta su una sorta di filiera industriale al servizio anche di altri territori del Paese. Questo è un dato molto interessante, perché di fatto in alcuni casi, che sono peraltro ben identificati e registrati, questa situazione determina o crea delle criticità. delle criticità ci sono, iniziando dalla Città metropolitana e dalla Provincia di Venezia, dove vengono identificati ben 240 siti contaminati e dove ci sono ben 439 siti da bonificare. Questa criticità viene fuori in Provincia di Verona, dove la situazione peggiore è in una zona, peraltro bellissima, della Valpolicella, nel Comune di Pescantina e nel sito cosiddetto di Ca' Filissine, dove si è venuta a creare una situazione drammatica dovuta alla continua perdita di una vecchia discarica, con inquinamento delle falde ed inquinamento dei suoli, in una situazione di grave abbandono da parte della società che gestiva tale impianto e che ha riversato la criticità sulle comunità. Questa criticità è registrata anche in provincia di Vicenza, in provincia di Treviso e in provincia di Rovigo, dove la centrale termoelettrica di Porto Tolle, che - come noi sappiamo - è una centrale di proprietà dell'ENEL ed è peraltro una delle più grandi d'Europa, per anni a funzionare mediante l'utilizzo di olio combustibile denso. Un'altra problematica che riguarda il Veneto è quella relativa alla questione dei fanghi di depurazione, che sono provenienti anche dal trattamento delle acque reflue urbane che pare siano prodotti largamente in eccesso rispetto all'effettiva esigenza del mercato e pertanto vengono spesso distribuiti in maniera illecita. Ora, in questa panoramica che ho voluto sintetizzare, seppur in una Regione che ha e vanta dei numeri e dei dati sicuramente significativi, sono venute fuori delle gravi irregolarità. Comunque, quello che bisogna sottolineare è che si tratta di irregolarità e talvolta di che comunque non vedono mai la presenza della criminalità organizzata. Situazione assolutamente diversa, invece, nell'altra relazione territoriale, quella sulla Regione Siciliana. dobbiamo registrare un ottimo lavoro compiuto dalla Commissione, una notevole quantità di dati acquisiti e una serie di approfondimenti assolutamente interessanti, da cui emerge che in Sicilia,

Assunzioni, clientele, nuovo precariato, mancanza di strategie, situazioni addirittura paradossali, in cui gli amministratori delle società di ambito, le cosiddette ATO, caratterizzate dal massimo delle clientele e della cattiva politica, sono stati, poi, nominati liquidatori delle stesse società,

una guida politica della Regione Siciliana poco autorevole, soprattutto in questi ultimi quattro anni, ritardi nell'esame delle richieste dei nuovi impianti o degli ampliamenti degli impianti già esistenti, ritardi che, peraltro, si registrano a discapito sia delle società pubbliche che di quelle private.

A tal fine si è prodotto un piano regionale dei rifiuti, che trovava attuazione in una posta di bilancio considerevole, circa 100 milioni di euro, che dovevano essere impiegati per la costruzione di tali impianti.

tra l'altro identificando commissioni di gara su nomina fiduciaria di natura esclusivamente politica, con componenti che oggi appaiono assolutamente imbarazzanti. Questo è il quadro in sintesi. Tutto questo ha creato e crea un'enorme confusione

non solo la cattiva politica e la cattiva burocrazia, ma in alcuni casi anche la criminalità organizzata. Questo è lo spaccato di quanto è avvenuto in Sicilia e di quanto continua ad avvenire,

Per arrivare alle conclusioni del mio intervento, mi rivolgo con un appello al Governo che vedo qui agitarsi in Aula: a mio avviso è arrivato il momento di una grande assunzione di responsabilità. di una grande assunzione di responsabilità. A dire la verità, l'abbiamo già registrata negli ultimi mesi con un cambio di passo e con un'attenzione elevata alla problematica e alla criticità siciliana, il che si deve alla guida politica del ministro Galletti e all'azione mirabile degli uffici (in particolare del direttore generale

incapacità e inadeguatezza, non può continuare a gestire il disastro. L'invito che allora rivolgo al Governo è di avere coraggio, perché questo chiedono oggi i siciliani nella stragrande maggioranza. Bisogna quindi procedere a

che individui quelle strategie che consentano di gestire questa fase di grande difficoltà e consentano alla Sicilia di uscire progressivamente da questa fase emergenziale, cercando di mantenere dritta la rotta verso un obiettivo che deve essere identificato e che allo stato non intravediamo, proprio per le politiche contraddittorie che hanno caratterizzato la gestione dell'intero settore dal 2002 a oggi. Questo è in sintesi il giudizio politico che diamo. Siamo grati, ancora una volta, alla Commissione per avere acquisito una quantità enorme di dati che oggi ci consentono di arrivare a queste conclusioni. Certamente, nell'ambito dei lavori in Commissione si poteva scendere più nel particolare,

che, a loro volta, si servono di fornitori non iscritti nelle *white list*. Sono tutte realtà che si sarebbe potuto approfondire, ma il dato che a noi oggi interessa è registrare la relazione nel suo valore complessivo e partire

Presidente, per un cittadino veneto leggere la relazione della Commissione è uno *shock*: una Regione è presa d'assedio dai veleni, con la pesante responsabilità della Giunta Zaia. Abbiamo 1.500 impianti di trattamento di rifiuti speciali, ma alcuni tra questi accettano illegalmente anche rifiuti pericolosi, che miscelano e smaltiscono falsificando i documenti. Anche gli impianti autorizzati per il trattamento non hanno una percentuale minima di recupero da rispettare, con il risultato che poi, magicamente, i veleni sono finiti nei sottofondi delle autostrade, come è successo nella Val d'Astico Sud: 150.000 metri cubi di veleni sono stati interrati e, nei terreni agricoli si trovano cianuri, arsenico, piombo e cromo. Ma fa gelare il sangue leggere nel documento che lo stesso rischio si potrà avere per la Val d'Astico Nord, come a dire che non si tratta di un fenomeno isolato, ma di un sistema. a chi servano davvero le grandi opere inutili, come l'autostrada Pedemontana che Zaia vuole, mentre (dati alla mano) non ha alcuna sostenibilità finanziaria, almeno al netto di possibili affari sporchi. Dimostrino il contrario, rendendo pubblici i dati finanziari. Troviamo poi l'assurdo dei fanghi di depurazione che sono in eccesso e, non trovando sbocchi di mercato, vengono sparsi nei terreni agricoli, spesso senza i trattamenti preliminari adeguati. In questo ambito operava la società Coimpo di Cà Emo, vicino ad Adria, dove il 22 settembre 2014 una reazione chimica tossica ha ucciso quattro lavoratori. Ci sono poi 485 siti contaminati e, tra questi siti, di società che operavano illegalmente, finché, scoperte e posti sotto sequestro gli impianti, sono fallite e i veleni sono là. Chi paga ora? Bisogna cambiare le regole: chi gestisce impianti e discariche non può solo presentare una fideiussione; mano a mano deve essere accantonato in anticipo anche il costo finale della bonifica. Pensate alla discarica di Pescantina, in provincia di Verona, gestita da Daneco Impianti in modo dissennato, al punto che il fondo si è rotto con fuoriuscita di enormi quantità di percolato. La società ha abbandonato il tutto e un piccolo Comune si ritrova ad affrontare Questi disastri, queste tragedie hanno un comune denominatore: la mancanza di controllo ed è a questo proposito che il lungo governo della Lega Nord ha precise responsabilità politiche, perché a capo della direzione tutela ambiente è stato posto Fabio Fior, condannato il 21 ottobre 2015 per abuso d'ufficio, falso, associazione per delinquere per reati ambientali e rinviato a giudizio per abuso d'ufficio, falso e peculato nel caso della riforestazione della discarica di Sant'Urbano, costata 5 milioni, ma non eseguita come dovuto. Nella relazione della Commissione si dice chiaramente che Fior ha potuto fare tutto ciò grazie alle coperture politiche di cui godeva. Questi disastri hanno un responsabile politico: Luca Zaia e la Lega Nord. Ma non sono gli unici: la ditta Miteni, nella Valle dell'Agno, da decenni produce sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) pericolose e associate a diabete, malattie della tiroide, aumentato rischio di infarto e *ictus* e, nei casi più gravi, cancro del rene, dei testicoli e altri tumori. Oggi, come ha denunciato il Movimento 5 Stelle, le falde sono inquinate in un'area enorme, che abbraccia più Province, nel bacino idrico più importante d'Europa e nei Comuni più contaminati abbiamo un aumento dal 10 al 30 per cento di queste malattie. Per risolvere la questione il ministro Galletti, anziché disporre misure urgenti, ha triplicato i valori di tollerabilità per queste sostanze: negli Stati Uniti vige la soglia di 70 microgrammi per litro, in Germania di 100 microgrammi per litro, in Italia erano 530 microgrammi, ma lui li ha portati a 1.500 microgrammi per litro. Questa è l'antipolitica che ci governa, criminale e miope se consideriamo che tutto ciò porterà enormi spese sanitarie nei prossimi anni; criminale e subdola se come sembra si stia dimostrando - sanno di scaricare questi costi sulle famiglie. Pensiamoci allora il 4 dicembre quando si voterà la riforma costituzionale: vale la pena di dare maggiori poteri a questo Governo? Vogliamo ancora un Parlamento alla sanità imposto da BCE, Commissione europea e Fondo monetario internazionale? Io dico no!

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti di cui faccio parte ha approfondito, attraverso l'acquisizione di documenti e informazioni assunte per mezzo di audizioni e sopralluoghi, la situazione attuale della Regione Sicilia in relazione al ciclo dei rifiuti. La risoluzione che oggi è all'esame di quest'Assemblea riguarda la relazione redatta dalla Commissione sulla situazione dei rifiuti in Sicilia, che è di estrema gravità. In Sicilia - come si evince molto chiaramente dalla relazione - è presente un diffuso illegalità connesso al ciclo dei rifiuti, che di fatto rappresenta un evidente ostacolo alla risoluzione dei problemi che attanagliano la Regione ormai da decenni. L'emergenza rifiuti della Sicilia parte da lontano, precisamente dal 1999, anno del primo commissariamento e anno in cui si tentò di porre fine al modello di smaltimento fondato su una discarica per ogni Comune, sostituendolo con un sistema di gestione conforme a quanto stabilito dal cosiddetto decreto Ronchi. Il risultato raggiunto fu ben diverso dalle aspettative. Se da un lato si raggiunse l'obiettivo di chiudere le piccole discariche, dall'altro queste vennero sostituite da quattro grandi discariche: Siculiana (Agrigento), Motta Sant'Anastasia (Catania), Mazzara Sant'Andrea (Messina) e Grotta San Giorgio (Catania), che ad oggi costituiscono la base del sistema di gestione dei rifiuti nella Regione Siciliana. Altro anno rilevante per spiegare la situazione di gravità in cui oggi versa la mia Regione è il 2002. Infatti, a partire da quell'anno vengono compiute alcune scelte scellerate: si decide di avviare la realizzazione di quattro megainceneritori e, contestualmente, di costituire gli ATO (ambiti territoriali ottimali). La strategia era chiara: da un lato, i Comuni non avrebbero dovuto più occuparsi della gestione dei rifiuti, giacché la Regione avrebbe affidato tale competenza agli dall'altro, la realizzazione dei quattro megainceneritori avrebbe consentito di chiudere il ciclo dei rifiuti della Sicilia. La costituzione degli ATO di fatto ha privato i Comuni delle proprie competenze generando una gravissima crisi finanziaria, derivante soprattutto dalla gestione poco trasparente e interamente in *deficit* svolta all'interno degli ATO, i quali come affermato anche nelle conclusioni della relazione - vengono utilizzati prevalentemente come strumento di consenso da parte della politica locale. La decisione di realizzare i quattro megainceneritori, che fu sospesa a seguito di alcune inchieste giudiziarie, ha provocato un totale disimpegno da parte delle amministrazioni comunali nel continuare la politica di raccolta differenziata, determinando un ulteriore peggioramento del sistema del ciclo dei rifiuti della Regione. Il quadro fin qui delineato è stato approfondito dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella precedente legislatura, conclusasi con la relazione del 2010. Come confermato anche dall'ANCI Sicilia nel corso dell'audizione del 3 novembre scorso presso la Commissione territorio, ambiente, beni ambientali del Senato, a partire dal 2010 la Regione Siciliana ha modificato la gestione del sistema integrato dei rifiuti, facendo cessare la gestione basata sui 27 ATO costituiti nel 2002 ed effettuando una nuova *governance* fondata su 10 ATO (uno per ogni Provincia e uno per le isole minori) e sulle società di regolamentazione, ossia le SRR (Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti). A partire dal 2012, è stata introdotta da parte della Regione una deroga al numero massimo di 10 ATO e, quindi, si è passati dai 10 agli attuali 18 ATO: uno per le Province di Enna, Siracusa, Ragusa e isole minori; due per le Province di Messina, Trapani, Agrigento e Caltanissetta; tre per le Province di Palermo A distanza di sei anni dalla riforma del 2010, si è arrivati al paradosso per cui gli ATO, diminuiti in un primo momento, non solo continuano a esistere, ma hanno anche duplicato le funzioni con la distinzione tra liquidatori e commissari di nomina regionale cui sono affidate funzioni di gestione. L'eredità lasciata dalle scelte effettuate a partire dal 2002, oggi, si riscontra nel fatto che molti territori siciliani sono invasi dai rifiuti e l'idea di portare i rifiuti fuori dalla Regione testimonia la totale crisi del sistema. Nell'estate appena trascorsa, poi, si è verificata l'esplosione dell'ennesima emergenza rifiuti, nel corso della quale sono state dettate da parte del governo regionale nuove disposizioni che, di fatto, hanno comportato per molti Comuni il conferimento della frazione indifferenziata dei rifiuti in discariche situate anche a diverse centinaia di chilometri di distanza da quelle in precedenza Dalla relazione redatta dalla Commissione, che riguarda la terza fase del commissariamento, dal 2013 al 2016, si evince chiaramente un quadro di corruzione molto grave e preoccupante, nel quale l'infiltrazione delle organizzazioni di stampo mafioso avviene in un secondo tempo e in maniera più subdola, ovvero nel noleggio a freddo,

in esercizio e attraverso la verifica delle tariffe da queste applicate. Inoltre, ha deciso di trasferire la competenza alla valutazione e al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) sulle discariche, dall'assessorato al territorio e all'ambiente all'assessorato all'energia e ai servizi di pubblica utilità. Qui è stato riscontrato un vero e proprio ostracismo da parte del dipartimento dell'ambiente, il quale avrebbe dovuto trasmettere la documentazione al dipartimento dell'acqua e dei rifiuti, a cui era stata affidata la nuova competenza in materia di istruttoria e rilascio dell'AIA. Da ciò è scaturito un quadro davvero allarmante, un quadro di corruzione di gravità devastante, consumato in un ufficio consumato in un ufficio cardine nel settore dei rifiuti, quale quello competente al rilascio delle autorizzazioni: fatti di una tale gravità da cui si può presumere una permanente deviazione delle funzioni pubbliche in favore di imprese private operanti nel settore dei rifiuti. Dalle attività della Commissione emergono altri tre dati allarmanti: il primo riguarda alcune società che, pur essendo coinvolte in indagini giudiziarie, continuano la loro opera di smaltimento dei rifiuti; iL secondo, sempre con riferimento alle infiltrazioni della criminalità organizzata, riguarda la creazione e il controllo di discariche discariche abusive sul territorio siciliano. Questi traffici di rifiuti sono stati resi possibili, evidentemente, dalla mancanza di adeguati controlli da parte degli organi preposti, preposti, non essendo pensabile che ingenti quantitativi di rifiuti possano circolare senza alcun tipo di controllo sul territorio siciliano, per poi giungere a destinazione in un sito non autorizzato. Il terzo dato di cui bisogna tener conto, signor Presidente, è che non esiste una vera concorrenza tra la *lobby* di chi vuole i megainceneritori e la *lobby* di chi ha la gestione delle discariche, perché in entrambi i casi sono presenti i medesimi gruppi, tant'è che nella relazione stessa si parla esplicitamente di «differenziazione dell'investimento illecito». La relazione fa emergere la necessità di effettuare una programmazione per la gestione del ciclo dei rifiuti, in modo da poter evitare il completo collasso del sistema in Sicilia. In conclusione va fatta una considerazione meritoria sull'operato della magistratura in Sicilia, laddove, anche dopo l'applicazione di misure cautelari reali su impianti e discariche di grandi dimensioni, ha assunto su di sé l'onere, congiuntamente agli organi amministrativi, di ricondurre la gestione degli impianti nella legalità. Signor Presidente, dal quadro appena descritto, emerge la mancanza di programmazione da parte della Regione Sicilia, che ha affrontato il problema relativo e ciò sicuramente non ha aiutato a risolvere il problema. Auspico, quindi, un intervento da parte del Governo - come peraltro è scritto nella risoluzione - affinché anche in Sicilia si possa arrivare a un quadro di programmazione e di legalità indispensabile per una gestione efficiente ed efficace del ciclo del ciclo dei rifiuti, in collaborazione con tutte le amministrazioni e gli enti interessati.*(Applausi 100, 200 e 301. Le proposte di risoluzione sono state distribuite. Ha la parola il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, dottoressa Degani, alla quale chiedo anche di esprimere il parere sulle proposte di risoluzione presentate.

il Gruppo dei Conservatori e Riformisti voterà contro la risoluzione Si tratta, per quanto ci riguarda, di una relazione che disegna un quadro allarmante quanto fuorviante di una Regione virtuosa, come riteniamo che sia la Regione Veneto. Come infatti conferma l'ultimo rapporto ISPRA sui rifiuti, nel Veneto si registra la più alta percentuale di raccolta differenziata, che è pari al 67,6 per cento, che ha come Comune capofila addirittura Treviso. La raccolta differenziata arriva addirittura all'81,9 per cento. Si tratta di un dato eccezionale che rappresenta il doppio circa della media nazionale, come rilevato da ISPRA, che si attesta al 45 È lontanissima da altre Regioni, tipo la Calabria e la Sicilia, con una raccolta differenziata abbondantemente sotto il 20 con oltre 60 milioni di presenze turistiche l'anno: un fattore, questo, che in qualche modo complica e appesantisce il sistema di raccolta e di gestione del rifiuto. Si arriva al paradosso di evidenziare come una criticità, un aspetto negativo la presenza in Veneto di ben 494 impianti pubblici di depurazione, di 1.500 impianti di trattamento dei rifiuti che utilizzano questi ultimi per produrre energia e recuperare materia prima, poiché questo - sostiene la relazione - è un numero elevato e, quindi, l'ARPA non potrebbe procedere ai controlli. La relazione, inoltre, non rende giustizia a una Regione che ha costituito un modello industriale sulla gestione dei rifiuti; un esempio di quella famosa economia circolare che ha addirittura anticipato in qualche fase le norme comunitarie. Il testo si basa su singoli casi negativi, effettuando una generalizzazione senza senso, in modo arbitrario per attaccare - come già detto - politicamente quella Regione. Si parla di illegalità diffusa, di controlli insufficienti, di carenza sanzionatoria, portando - ad esempio - come cartina di tornasole, la vicenda di un unico funzionario del Veneto che è stato inquisito.

Ad oggi il risultato che ci troviamo in Sicilia è che le discariche comunali sono chiuse, ma quattro discariche più grandi hanno preso il loro posto - e dico ben quattro - per la maggior parte gestite da soggetti privati da soggetti privati con autorizzazioni a dir poco discutibili. Addirittura si parla di 27 ATO; e di queste ultime si vede in maniera molto netta che vengono utilizzate più per assunzioni clientelari. Quello che emerge dalla relazione è che ci troviamo di fronte ad un sistema di illegalità illegalità diffusa, dove trovano terreno fertile associazioni criminali e clientele, fin dentro le istituzioni siciliane, dove manca a tutt'oggi una seria programmazione, tanto che il Ministero dell'ambiente ha voluto continuare nella gestione commissariale. Insomma, quello che abbiamo potuto osservare è che emergono soltanto opacità e mancanza di controlli, infiltrazioni di un sistema criminale che passa dall'amministrazione regionale ai Comuni che, a fronte di bandi - per esempio - per l'assegnazione del servizio raccolta rifiuti, vedono partecipare una sola impresa, come se ci fosse stata una spartizione a tavolino del lavoro dei Comuni che bandiscono La stessa procura di Palermo conferma la deviazione delle funzioni pubbliche in favore di privati, in particolare per il rilascio dell'AIA rispetto alle discariche che prima abbiamo citato. E molte sono le criticità che come Commissione abbiamo in qualche modo fatto nostre e raccolto. Anche l'ANAC individua tutte le criticità che noi abbiamo rilevato: conflitto di interessi, incarichi professionali assegnati senza qualifica, progressione di carriere legata non alla capacità dei funzionari pubblici,

Presidente, colleghi, onorevole Sottosegretario, il Gruppo Lega Nord e Autonomie voterà contro la relazione territoriale sulla Regione Veneto proposta dalla Commissione d'inchiesta. Riteniamo che questa volta la Commissione sia andata oltre i confini dell'obiettività e dell'imparzialità che la dovrebbero caratterizzare, trasformando piuttosto il documento in un attacco politico contro la Regione Veneto e il suo Governo. Si tratta di una relazione impostata male, che pecca di superficialità, che ricorre talvolta anche a toni dispregiativi, che arriva a confondere il lettore in 455 pagine di testo e che prende come esempio la Regione più virtuosa in materia di gestione di rifiuti - e non solo rifiuti solidi urbani - e la presenta come il peggior

capofila la provincia di Treviso che, nel 2014, ha superato l'80 per cento. Si tratta di percentuali che raddoppiano quasi il dato nazionale dell'ultimo rapporto ISPRA, che si attesta al 45,2 per cento, contro dati regionali vergognosi come il 18,6 della Calabria e il 12,5 della Sicilia, Regione quest'ultima oggetto oggi dell'altra relazione al nostro esame. Non dimentichiamoci, inoltre, che la Regione Veneto presenta un PIL tra i più elevati del Paese e registra oltre 60 milioni di presenze turistiche annue che - lo sappiamo benissimo - impattano negativamente sulla raccolta differenziata. Sono 494 gli impianti pubblici di depurazione e 1.500 gli impianti di trattamento che utilizzano i rifiuti per il recupero di energia e di materia. Il paradosso è che la relazione della Commissione d'inchiesta critica questo elevato numero di impianti poiché impedirebbe all'ARPA di effettuare controlli efficaci. Si tratta di forzature lampanti, di una palese esagerazione. La relazione non rende giustizia ad una Regione che, negli anni, ha costituito l'esempio della struttura imprenditoriale nella gestione dei rifiuti verso un'economia circolare che ha anticipato anche le norme comunitarie; un'economia circolare oggetto, questa settimana, anche della fiera Ecomondo di Rimini, in cui molti Presidenti di Regioni e amministratori locali parlano a vanvera, perché lontani anni luce dall'averla minimamente impostata e perseguita sul proprio territorio. Il testo si basa su singoli casi per attaccare politicamente la Regione utilizzando espressioni inappropriate. Si parla di «contesto di illegalità diffusa, controlli insufficienti e carenze sanzionatorie» di cui costituisce la cartina di tornasole la vicenda di un dirigente regionale. Si è impiegato, cioè, un tono dispregiativo per descrivere la vicenda di un funzionario - certamente grave, ma isolata e sulla quale, caro collega Endrizzi, il presidente Zaia ha da subito collaborato con la procura della della Repubblica - per rappresentare la Regione Veneto come un contesto di illegalità diffusa. Stiamo parlando davvero della Regione Veneto in questa relazione, oppure della Sicilia, della Calabria o della Campania? Si avanzano poi affermazioni di influenza dell'organo politico sulle valutazioni ambientali degli impianti e si elencano le distorsioni e le elusioni delle norme che normalmente avvengono sul mercato presentandole come «il vero problema del Veneto». In merito alla vicenda Miteni e sull'inquinamento da PFAS, caro collega Endrizzi, informati e scoprirai che, in assenza dei limiti tabellari che lo Stato non ha imposto, la Regione ha avuto un approccio al problema che è stato molto apprezzato. In merito all'utilizzo di scorie nel sottofondo autostradale della Valdastico, sottolineiamo che si tratta di una pratica comunemente utilizzata e permessa dalla normativa comunitaria vigente. La relazione della Commissione, comunque, non si limita all'evidenziazione dei superamenti del caso specifico - sul quale, prima di criticare, occorrerebbe controllare 1'eventuale compatibilità con il fondo naturale - ma, alla pagina 28, estende la critica anche alle norme dei requisiti della miscelazione e della cessazione della qualifica di rifiuto, previste dall'Unione europea e regolarmente approvate dal Parlamento, e sulla validità delle metodiche da utilizzare per l'esecuzione del test di cessione ai fini della verifica del rispetto dei requisiti di compatibilità ambientale. queste ultime, rimaste invariate già dal 1998, ai sensi del decreto ministeriale del 5 febbraio 1998 di attuazione del decreto Ronchi. Pertanto, le critiche della relazione della Commissione si estendono anche alle modalità democratiche di approvazione delle leggi, probabilmente perché l'estensore della relazione non era d'accordo al momento della votazione. In merito all'esportazione dei RAEE a Hong Kong, in India e in Malesia, la relazione non fa alcun cenno sul fatto che si tratta di un fenomeno mondiale e che, accanto a Venezia, anche altri porti come Bari, Napoli, Ancona, Civitavecchia, Salerno, Taranto, La Spezia, Pozzallo, Genova, Gioia Tauro, Livorno e Catania sono coinvolti in inchieste varie per l'esportazione di rifiuti e che il transito di RAEE attraverso l'Italia avviene, principalmente, perché il nostro Paese viene considerato quello con la legislazione meno rigida in materia. Grave infine - e lo voglio qui ancora denunciare - è la pubblicazione su «ilfattoquotidiano.it» dello scorso 21 maggio 2016 di notizie riservate, evidentemente fatte uscire sotto banco dal palazzo, riguardanti la relazione ancora a quel momento non approvata dalla Commissione d'inchiesta. Sfruttando solo alcune parti della relazione, è stato evidente lo scopo di denigrare e diffamare una Regione

La relazione mette in evidenza tutte, molte, troppe problematiche, criticità e vere patologie che da anni hanno compromesso il settore della gestione dei rifiuti nella Regione. Illegalità diffuse e radicate hanno ostacolato la risoluzione dei problemi,

è - colleghi - la base per superare l'emergenza e rientrare nella gestione ordinaria ed evitare le gare in deroga. La previsione di quattro mega inceneritori, mai realizzati, che ha favorito lo smaltimento in discariche; le carenze della raccolta differenziata, che si attesta al solo 12,5 per cento, contro - lo ripeto - il 67,6 per cento del Veneto; l'assegnazione di ingenti fondi pubblici a società che hanno sottoscritto patti di integrità con la Regione, ma che non risultano iscritte nelle *white list* delle prefetture, dimostrano l'inefficienza delle autorità di governo e di controllo. A ciò si aggiunge la gravissima crisi finanziaria conseguente alla deficitaria e non trasparente gestione dei ventisette ATO, che sono stati uno strumento che rispondeva a una logica clientelare in mano alla politica per il controllo del consenso. In particolare, alcune scelte decisionali hanno penalizzato le imprese di tutto il Paese, che hanno lavorato nel settore dei rifiuti della Regione e che non riescono ancora a recuperare i propri crediti. E, fra queste, molte moriranno per eccesso di credito non riscosso. E che dire delle nomine in posti cruciali per la gestione dei rifiuti di soggetti incompetenti e completamente estranei del settore. Restano ancora da approfondire le ipotesi di affare sui quattro inceneritori, la cui mancata realizzazione sembra sia stata frutto di accordi tra il mondo politico-amministrativo, il mondo economico e le associazioni criminali per poter - da un lato - favorire e proseguire le attività di smaltimento in discariche derivate e - dall'altro - per creare le condizioni per poter trasportare i rifiuti fuori regione. Purtroppo, la stratificazione normativa e il macchinoso apparato burocratico hanno permesso a funzionari corrotti di rilasciare facili provvedimenti autorizzativi che agevolano gli imprenditori alimentando un sistema corrotto. Come evidenziato dalla Commissione d'inchiesta, l'infiltrazione della criminalità organizzata di stampo mafioso nel settore dei rifiuti, a tutti i livelli, avviene prevalentemente approfittando delle carenze amministrative, attraverso il controllo degli appalti e delle attività accessorie al settore dei rifiuti vero e proprio, quali il trasporto, la manutenzione dei mezzi e le forniture. In conclusione, voglio stigmatizzare il comportamento ambiguo del Governo e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, di fronte all'emergenza rifiuti dell'Isola, se da una parte non ha rinnovato il commissariamento della Regione, dall'altra ha concesso al presidente Crocetta la possibilità di firmare una nuova ordinanza contenente una serie di deroghe sia sul trattamento dei rifiuti indifferenziati, sia sulle autorizzazioni per lo smaltimento in discarica, sia, infine, sulla costruzione degli impianti e l'adeguamento del piano regionale. È pertanto opportuna la relazione della Commissione d'inchiesta, che si auspica possa essere di impulso

delle comunità che sono diventate punto di riferimento di altri Comuni del Paese,

è forse legato al fatto che tante piccole e medie imprese, nel momento della crisi e della difficoltà economica, hanno fatto una scelta di guadagni più semplici e facili, cercando soluzioni che permettessero lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e speciali attraverso

discariche private. Tali vicende ci dicono quanto i controlli regionali siano inesistenti e sono la prova provata di quanto siano ramificati in questo settore la corruzione e il rapporto con la criminalità organizzata. Pensiamo soltanto alle convenzioni stipulate per la costruzione dei quattro megaimpianti di incenerimento, che non sono state revocate neanche dopo l'intervento della Commissione europea. Queste vicende che hanno caratterizzato e contrassegnato la questione degli inceneritori e anche quelle relative alle autorizzazioni ci dicono di un *modus operandi* operandi* assolutamente illegale, illegittimo e per buona parte criminale. Quindi, oltre che l'ambiente, è inquinato l'intero sistema di gestione dei rifiuti della Regione,

mista anche alla mancanza di volontà politica e amministrativa, di predisporre una seria programmazione del ciclo integrato dei rifiuti. rifiuti. La mancanza di programmazione corrisponde quindi a un approccio basato costantemente sull'emergenza, sulla contingenza e sull'approssimazione. Non casualmente, non è soltanto incapacità gestionale,

illegale di tutta la gestione. Si continua a gestire la raccolta differenziata, il trattamento dei rifiuti indifferenziati, le autorizzazioni all'abbancamento in discarica, l'adeguamento del piano regionale e persino la questione degli inceneritori attraverso una serie di provvedimenti derogatori, che escludono - tra l'altro - dai momenti decisionali quasi tutte le comunità locali. Quindi la Sicilia è emblematica del fallimento totale del sistema commissariale della gestione emergenziale del ciclo dei rifiuti.

plateali e insopportabili, a danno dei cittadini e dell'ambiente. Anche su questo tema noi apprezziamo il lavoro fatto dalla Commissione e daremo il nostro voto favorevole

e la criticità della gestione commissariale, nonostante la gestione di questo sito sia iniziata addirittura nel 2007. Ma evidentemente è proprio questo che non funziona, questo tipo e questa modalità di gestione. La relazione ci dice che la situazione della contaminazione risulta irrisolta, che si sovrappongono attività diverse e che il potenziale impatto - questo è l'elemento più preoccupante - della contaminazione sulle

Signora Presidente, in un breve intervento confermo il voto favorevole del Gruppo parlamentare al quale appartengo sulle proposte di risoluzione oggi all'esame del Senato.

In Sicilia dobbiamo registrare un sistema le cui colpe e responsabilità non sono obiettivamente ascrivibili soltanto a chi oggi ha la guida politica della Regione;

del presidente Crocetta, che oggi è alla guida politica della Regione, è di non aver assunto in prima persona, fin dal primo momento, la diretta responsabilità dell'intero comparto,

mi permetto di dissentire totalmente dall'intervento che ho ascoltato, esplicitato dal collega della Lega perché l'unico elemento positivo è il tentativo del Ministero dell'ambiente, che da un anno a questa parte, attraverso il concerto preventivo, ha determinato delle ordinanze assolutamente precise e ristrette che non consentono alcuna discrezionalità

della raccolta differenziata e la diminuzione dei volumi trattati. Questi sono dati innegabili. Sono convinto che questa direzione debba vedere - come ho detto nel mio intervento precedente - una Grazie,

responsabili, in particolare le procure della Repubblica, che possono istituzionalmente intervenire in questo settore, da lì possano trarre una serie di valutazioni assolutamente dirimenti.

del senatore Compagnone, anche se ne condividiamo le premesse e le considerazioni, ma non la richiesta al Governo, che esplicitamente chiede di provvedere a un commissariamento della Regione Siciliana.

c'è stata una variazione che a mio giudizio è sostanziale, perché tende a dare una visione diversa dell'opportunità e delle finalità di questa ordinanza, che, nella prima versione, era vista come un provvedimento derogatorio, o comunque di urgenza che non si nella linea dell'ordinario. Viene stralciata tutta la parte che fa riferimento all'urgenza e ribadito che, a differenza del passato, l'ordinanza, chissà per quali motivi, riuscirà a risolvere i problemi, e non è il mondo dei sogni di cui ho parlato prima, ma sicuramente un documento realistico. Nonostante questo voteremo a favore della risoluzione ciò che conta è il lavoro che la Commissione ha fatto sulla relazione e l'appello che viene rivolto al Governo è di adottare provvedimenti anche legislativi al riguardo. Gli studi della Commissione anche a questo servono, a riflettere sulle necessità normative, su quanto occorre ed è necessario mutare nelle nostre leggi. La Commissione ha lavorato bene, come hanno lavorato bene le Commissioni delle delle precedenti legislature, e ha messo nero su bianco quelli che ad ogni evidenza sono i grandi problemi del nostro Paese. Eppure, sembra

Per quanto riguarda il Veneto si evince un'elevatissima contaminazione ambientale, di tutte le matrici, in aree densamente abitate. Da ciò si deduce, come per tante altre relazioni, la necessità di un maggiore controllo, laddove questa legislatura sta andando nella direzione di un minore controllo che viene venduto come semplificazione. Occorre un maggiore controllo degli impianti e dare al sistema delle agenzie ambientali un maggior sostegno finanziario, strumentale e umano per poter fare i controlli necessari. Bisogna creare una forza di polizia ambientale nazionale, (abbiamo visto come siamo andati a finire con il Corpo forestale dello Stato). I 1.500 impianti di trattamento rifiuti speciali che sono nella Regione Veneto hanno evidenziato come, anche lì, sia vastissimo l'uso della falsificazione il classico giro di bolla che ben conosciamo noi della Regione Campania. Non ha importanza che qui non ci siano infiltrazioni camorristiche, della 'ndrangheta

che in pratica sono rifiuti vengono poi trattati come non rifiuti. Nella Regione Veneto si contano 485 siti contaminati per gestioni illecite di rifiuti speciali e pericolosi; però, quando poi le aziende che hanno che hanno gestito così male questi siti vengono sequestrate, queste falliscono e quindi ci troviamo nella condizione di non poter provvedere alle bonifiche perché gli enti territoriali sono sprovvisti delle risorse necessarie. Per questo, come già ho ribadito in altre occasioni, è necessario stabilire in modo netto e chiaro per tutte le attività impattanti un accantonamento obbligatorio, vincolato - direi blindato - di somme che siano proporzionali al tipo di produzioni e al rischio stimato di contaminazione finalizzate esclusivamente al ripristino ambientale e alla bonifica, anche soltanto in fase di dismissione. Mi riferisco ad un fondo di cui bisogna dare contezza e certezza anche anche semplicemente durante le richieste di autorizzazione integrata ambientale, di rinnovo e di ampliamento e - lo ripeto - per tutte le attività produttive impattanti.

ma evidenziano l'aumento della malagestione, dell'inquinamento ambientale e dell'infiltrazione malavitosa. Lo dicevamo per strada in Campania prima di venire in questa sede lo ribadiamo ancora, eppure si continuano a varare provvedimenti urgenti.

la criminalità (organizzata o no, con le infiltrazioni mafiose o no) è il vero cancro da combattere; tuttavia, senza una vera riforma del sistema giudiziario, che questo Governo si ostina a ritardare, a non voler fare, a non far passare, non ne usciremo mai. È vero che l'anno scorso è stata approvata con grande difficoltà la legge n. 68 che sta dando buoni risultati, ma da sola non può bastare. È necessaria l'istituzione del DASPO per i condannati, cioè la preclusione a qualunque rapporto

al rinvio a giudizio, che almeno venga fermata alla condanna di primo grado, anche per evitare che i tribunali vengano affollati da ricorsi da ricorsi soltanto strumentali a giungere alla prescrizione (sappiamo che nel sistema italiano il secondo e terzo grado non possono essere peggiorativi per il condannato appellante). Bisogna potenziare il reato di autoriciclaggio, il reato di voto di scambio politico-mafioso

Grazie,

di legalità compiuta nell'ambito del riciclo dei rifiuti e quindi nella gestione complessiva del ciclo dei rifiuti, per arrivare a quell'economia circolare che dovrebbe diventare la nostra forma

che ha prodotto quanto di peggio dal punto di vista degli sversamenti e delle discariche. La chimica è un settore pesante che ha lasciato un sito contaminato che le autorità locali non sono riuscite finora a mettere in piena sicurezza, seppure vi siano stati dei passi in avanti. Ma anche su questo aspetto la relazione intende mettere in evidenza le lacune che vi sono state nel corso di questi anni e in qualche caso di questi decenni nella politica locale, nella politica nazionale e anche nei rapporti tra privati, in particolare tra imprese e politica.

sta lavorando bene - è di recuperare il tempo perduto, arrivando a un'individuazione rapida delle azioni da compiere per la definitiva messa in sicurezza e bonifica di un'area che, voglio ricordare, riguarda 11 Comuni, quindi è vastissima.

chi era il gestore politico, e lo dimostrano le risoluzioni che abbiamo già approvato in Senato. Mi spiace che per la parte riguardante il Veneto si sia fatta un'eccezione; poi spiegherò che questa eccezione non ha alcun senso di esistere.

andando in quel territorio e anche audendo all'interno della Commissione i sindaci coraggiosi di questo territorio ed alcuni amministratori regionali sensibili. Ebbene, questa infiltrazione mafiosa ha reso possibile la realizzazione di discariche abusive di proporzioni sistemiche e vastissime, prive spesso di qualsiasi autorizzazione e quasi sempre nell'immediata disponibilità e proprietà delle cosche. Traffico di rifiuti di ampie dimensioni, mancati controlli da parte degli organi preposti, minacce, noleggi a freddo, subappalti, assunzioni improprie,

dell'ARPA locale, determinata da carenza di organico e dall'impossibilità spesso di poter procedere. Il secondo elemento è un'amministrazione pubblica assolutamente assente, quando non connivente nel settore dei rifiuti, in particolare con le aziende che si erano inserite in questo settore, ma con l'unico scopo di fare *business*,

perché dovremmo spendere 65 milioni di euro, come Ministero, per la messa in sicurezza e la bonifica di una delle peggiori discariche d'Italia, con 30 metri di percolato,

degli stessi di quote del corrispettivo versato dalle aziende che conferiscono i rifiuti, in modo da costruire un fondo di riserva, che affronti le successive operazioni, in garanzia per i cittadini e le comunità locali, di messa in sicurezza dei siti inquinanti. Ancora, come diceva bene la collega Nugnes, per evitare la proliferazione e la prosecuzione di comportamenti sistematicamente illegittimi, che abbiamo visto essere di grande pericolosità sociale e sanitaria, occorre inserire all'interno della normativa sugli ecoreati il sequestro per equivalente, ritenuto dalle Forze dell'ordine, dalla magistratura, nonché dai sindaci uno strumento utile, che va ad implementare la normativa recentemente

Procediamo ora con la votazione delle proposte di risoluzione che saranno poste ai voti nell'ordine di presentazione relativo a ciascun documento.

a precisare le finalità generali della legge. Esiste anche un contesto giuridico internazionale e comunitario all'interno del quale dovrebbe essere collocato, giustamente, il nostro sistema delle aree protette e dunque anche il disegno di legge, con particolare riferimento - e questo è il senso dell'emendamento - agli atti relativi in materia di tutela della biodiversità e della conservazione degli *habitat* naturali

assolutamente fondamentale fare in modo che si possa dar vita ad un programma triennale relativo alle aree protette,

temi all'attenzione di tutti coloro che si occupano del sistema delle aree protette. Infatti soltanto una prospettiva di rilancio degli investimenti la conservazione e la tutela degli *habitat* naturali del sistema delle aree protette potrebbe assicurare un adeguato rilancio del sistema dei parchi e delle aree protette

un aumento delle accise sulle materie prime energetiche a più alto impatto in termini di emissioni climalteranti. Questo è un emendamento che consideriamo particolarmente importante perché

solo allo Stato centrale - al fine di evitare, per i tratti di mare contigui alle aree protette regionali, una doppia gestione e doppi oneri a gravare sul bilancio dello Stato.

con le seguenti: «Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente» per attualizzare il disegno di legge dopo la recente entrata in vigore della legge 28 giugno 2016, n. 132, relativa al riordino del sistema nazionale a rete delle agenzie ambientali.

in fase di discussione della modifica del testo unico sui parchi, avevano sollecitato sia il Ministero che le Regioni a convocare questa terza conferenza al fine di discutere di queste variazioni ma questo non è stato accordato. visto che il provvedimento passerà in questi giorni, chiediamo che essa sia convocata e che si svolga, per mettere a punto tutte le problematiche e tutti gli obiettivi futuri per quanto riguarda le nostre aree protette.

per l'avvio, su iniziativa di giovani di età inferiore a 40 anni, di attività economiche in alcuni settori che possono innescare sinergie virtuose per la gestione delle aree protette e la promozione delle attività sostenibili. Esso riguarda anche specificamente i Comuni il cui territorio è inserito, integralmente o in parte, all'interno del sistema delle aree protette. La copertura che avevamo individuato (e su cui

per cento delle *royalty* derivanti dalle attività di estrazione degli idrocarburi in mare, come peraltro era stato già richiesto dalla risoluzione approvata dalla Commissione ambiente del Senato addirittura nel marzo 2014.

non prevede altro che, qualora il territorio del parco o della riserva naturale ricomprenda siti militari, aree individuate per esercitazioni e/o poligoni di tiro,

l'emendamento possa essere un segnale forte a difesa del territorio e null'altro: non ha nessun'altra finalità.

così restrittiva mi lascia parecchio perplesso, non conoscendone - ripeto - nemmeno le motivazioni, visto e considerato che stiamo parlando di nuove disposizioni a tutela delle aree protette.

che devono essere abbandonate al loro destino, ditelo chiaramente. In caso contrario, credo che il minimo possa essere l'accoglimento di un

4.103 chiediamo che, in ordine alla nomina del Presidente del parco, l'intesa debba essere cercata non solo con riferimento alle Regioni, ma anche alla comunità del parco, che riteniamo debba essere adeguatamente rappresentata.

un po' un tornare indietro, al dettato della vecchia legge n. 394 del 1991, in cui viene ribadito che le persone che faranno parte del consiglio direttivo verranno scelte tra coloro che hanno particolari qualificazioni per le attività in materia di conservazione della natura, gestione delle aree protette, diritto amministrativo e ambientale e non soltanto quota parte di esse. Si propone altresì che vedeva sparire il membro di ISPRA nella conformazione minore a vantaggio del rappresentante degli agricoltori, ossia di un imprenditore. Invito quindi l'Assemblea a votare a

tra i membri designati dalla comunità del parco e i rappresentanti di interessi più generali e più diffusi, nonché la qualificazione

indicando una specializzazione del settore: non basta essere stato un bravo dirigente genericamente, in un altro settore della pubblica amministrazione.

un'indicazione molto chiara e precisa dei requisiti e delle competenze gestionali specifiche nel campo.

una cosa abbastanza strana e singolare. Nell'emendamento si prevedono infatti delle figure che non vanno ad incidere più di altre dal punto di vista economico.

intervengo molto brevemente sull'ordine dei lavori. Non intendo minimamente mettere in discussione il suo operato, ma vorrei richiamare l'attenzione sulla procedura assolutamente inusuale che è stata utilizzata a proposito dei due emendamenti Non è mai stato possibile e sarebbe un precedente pericolosissimo per i lavori dell'Aula - perché l'opposizione potrebbe profittarne in maniera anche eccessiva sottoporre ad un nuovo giudizio della Commissione bilancio un emendamento già dichiarato improcedibile,

parere della Commissione ed anche la stessa procedura dell'articolo 100, che lei ha invocato, è prevista solo ed esclusivamente in presenza di modifiche ai testi già presentati in Aula. Pertanto, faccio appello anche alla sensibilità del relatore affinché non ceda a questa tentazione che potrebbe introdurre un precedente pericolosissimo. D'altronde, i presentatori hanno la facoltà di richiederne comunque la votazione

c'era la dichiarazione di alcuni senatori che ricordavano che il parere era stato diversamente formulato e, quindi, c'è stata una verifica dell'esatta dell'esatta trascrizione del parere. Sul secondo, siccome c'è stata una sollecitazione forte del relatore, per tentare di rendere più collaborativo il rapporto tra il relatore, il Governo ed altri senatori, mi è sembrato opportuno consultare il Presidente della Commissione bilancio, senza che questo costituisca una *diminutio* della forza del parere *ex* articolo 81.

per confermare la sequenzialità del provvedimento, propongo che prima di votare gli emendamenti all'articolo 4 si ritorni ad affrontare, concludendolo, l'articolo 2, posto che non rimane nulla che osti a trattare gli emendamenti presentati all'articolo 2. Il presidente Tonini si è espresso perché aveva la parola. Credo che per l'ordine dei lavori sia meglio concludere un articolo e non interrompere anche l'articolo 4, ritornare indietro e poi in avanti. Quindi, adesso concludiamo l'articolo 4 e, poi, "chiuderemo" anche l'articolo 2.

Noi siamo liberali e riteniamo che, nella loro autonomia, coloro che amministrano la cosa pubblica,

così rischiando di escludere la libertà di azione in ciò che non è previsto dalla legge. Secondo me, che l'ente parco possa fare convenzioni con altri enti

- se stabiliamo per legge che queste cose si possono fare, mettiamo a rischio altre eventuali attività che, in corso d'opera, l'ente parco voglia mettere in piedi, ma che, non essendo previste dalla legge secondo un'interpretazione dei rapporti sociali che non ci è assolutamente confacente, possa eventualmente avere delle remore a fare.

le questioni che avevamo sollevato, in particolare quella sulle competenze specifiche, sia in ordine alla scelta e alle caratteristiche del presidente, sia

non dovrebbero forse già avere occupato il 100 per cento del loro tempo. Invece qui si stanno producendo delle modifiche per cui dovranno fare i senatori, i presidenti degli enti di area vasta, i presidenti delle aree metropolitane e adesso devono anche entrare all'interno dei consigli direttivi dei parchi. Io onestamente comincio ad avere - non è una battuta - una serie di perplessità; sarà forse perché vengono date sempre meno risorse agli enti locali e quindi evidentemente forse si pensa di compensarli con altro. Ma credo che non faccia bene né ai sindaci, né, in questo caso, alla gestione dei parchi. La nostra proposta, come quella di altri senatori, tendeva a ristabilire in qualche modo un equilibrio tra i rappresentanti della comunità del parco - per la verità io avrei previsto anche un rafforzamento della comunità, non tanto nella nomina, ma proprio nei poteri stessi - e contemporaneamente cercava di fare in modo che i parchi non subissero, come invece in questo modo avviene, una deriva verso una *governance* che rischia di risentire sempre di più di interessi localistici. Le competenze e la *mission* che hanno i parchi e le aree protette, e quindi i consigli direttivi, è evidentemente quella di farsi carico di interessi molto generali e diffusi, quali appunto la tutela degli *habitat* naturali e la conservazione della natura. Perfino nella vostra riforma della Costituzione - che noi, com'è noto, combattiamo e combatteremo

Signora Presidente, con questo intervento di fine seduta continuo oggi al Senato una staffetta con cui, assieme a tante senatrici e tanti senatori, ricordiamo ogni donna che viene uccisa per mano di un uomo, a cui è, o è stata, legata da una relazione amorosa. Lo faremo fino a che sarà necessario ricordare al Parlamento e al nostro Paese l'urgenza di arginare la violenza nei confronti delle donne. Violenza che si manifesta in tanti modi: la violenza fisica, verbale, psicologica ed ultima ma non meno aberrante, la violenza economica.

Il 3 novembre a Bitonto, in provincia di Bari, Mariagrazia Cutrone, di ventinove anni è stata uccisa a coltellate dal marito, che poi ha tentato il suicidio. La sera prima Mariagrazia, madre di tre figli di tre, cinque e sette anni, aveva chiesto aiuto ai carabinieri che, dopo un chiarimento fra i coniugi, avevano redarguito verbalmente il marito e li avevano rimandati a casa. Il 4 novembre è stata la volta di Viktoria Shovkoplyas, cinquantaquattro anni, morta a Ottaviano, in provincia di Napoli, a seguito di una violenta spinta ricevuta dal suo compagno, durante un litigio: le ha provocato una grave ferita alla testa. L'uomo non ha chiamato subito i soccorsi dopo l'accaduto ed è ora accusato di omicidio preterintenzionale.

trent'anni di carcere nei confronti del compagno che aveva confessato di averla ammazzata. Salgono così a 24 le donne che ricordiamo in questa staffetta, iniziata solo il 30 giugno. Contiamo, più o meno, cento decessi dall'inizio del 2016. invece sventato a Magenta, grazie all'intervento dei carabinieri (chiamati dalla donna che non ha accettato di uscire di casa per un ultimo chiarimento), un tentativo di femminicidio di una donna di quarantun anni ad opera del suo ex fidanzato. L'uomo si era infatti presentato sotto casa della sua ex con un coltello e una bottiglietta di acido muriatico, coi quali - come ha ammesso - aveva l'intenzione di colpirla. Già denunciato per *stalking*, l'uomo è ora in carcere con l'accusa di atti persecutori. Come anche questi casi dimostrano, il femminicidio è quasi sempre l'estremo risultato di una serie di comportamenti violenti di lunga data. Il femminicidio è, in ultima analisi, la reazione, violenta e vigliacca, all'incapacità di rispettare la libertà delle donne. Con la legge n. 119 del 2013 di contrasto alla violenza di genere, che questo Parlamento ha approvato in attuazione della Convenzione di Istanbul, il nostro Paese ha riconosciuto la violenza sulle donne come violazione dei diritti umani e discriminazione di genere. Ha riconosciuto che la violenza sulle donne è un fenomeno sociale, un fenomeno che ha radici pubbliche e non private. La violenza di genere e i soprusi sulle donne, sono alimentate dalla cultura patriarcale fortemente stereotipata e radicata nella nostra società. Questo sistema discriminatorio, man mano, si sta scardinando: gli uomini riconoscono e rispettano sempre di più le donne come professioniste ed esseri umani liberi e le donne acquistano sempre di più consapevolezza della propria indipendenza. Questo fenomeno si può prevenire, intervenendo sui fattori che lo determinano, applicabili in molteplici ambiti: giuridico, lavorativo ed educativo. A tal fine è stato proposto e approvato un piano contro la violenza sulle donne. Nel frattempo sono stati rafforzati strumenti di protezione per garantire maggiore sicurezza alle donne minacciate. Bisogna però continuare a monitorare che queste misure funzionino e che il piano sia attuato. Ma per rafforzare le garanzie e tutele a difesa delle donne, dobbiamo domandarci: come mai la rete di protezione che ha salvato la donna di Magenta non ha invece funzionato nel caso di Mariagrazia a Bari? Qualche settimana fa, nella città di cui mi onoro di essere stato sindaco, si è discusso approfonditamente di questo tema, e approfitto per ringraziare la vice presidente del Senato Valeria Fedeli che è venuta a dibattere assieme a tante giovani donne e giovani uomini su questo tema. Noi riproponiamo con convinzione il nostro appello. Un appello alla Ministra per le pari opportunità e al Governo tutto: la cabina di regia, che si è riunita per la prima volta l'8 settembre scorso, monitori l'applicazione, i pregi e i limiti della legge n. e soprattutto dia piena e accurata attuazione al piano contro la violenza. Un appello ai *media*: che assumano finalmente il ruolo di educatori della società, promuovendo un linguaggio che rifletta una società paritaria e giusta, descrivendo la reale portata del femminicidio, come fenomeno sociale, e non come sporadico evento attinente alla vita di coppia; valorizzino, veramente, il ruolo della donna nella compagine sociale. Concludendo, un appello al Paese, uomini, soprattutto, e donne: sono 160 le donne uccise ogni anno. Non possiamo più accettare questa mattanza.

Presidente, colleghi, il 25 maggio scorso la Commissione ambiente ha approvato il Documento

La necessità della Commissione d'inchiesta è dimostrata non solo dai vari illeciti che hanno contraddistinto il processo di ricostruzione in questi anni, molti peraltro già oggetto di inchieste da parte della magistratura, ma anche dalle lesioni subite da alcune abitazioni appena appena ricostruite e recentemente restituite ai proprietari, a seguito delle scosse di terremoto del 24 agosto. Danneggiamenti sono stati registrati in alcuni condomini di via Amiternum e a Cansatessa e Santa Maria di Farfa, sebbene giudicati non pericolosi dai tecnici e dai Vigili del fuoco che hanno effettuato i sopralluoghi; invece, per gli edifici di edilizia residenziale pubblica di San Gregorio è stato ordinato lo sgombero di molte famiglie, dopo averle fatte vivere per sette anni

l'ennesima inchiesta. Questi ultimi sviluppi impongono ancor di più l'apertura di rigorosi accertamenti circa l'esemplarità di gran parte dei lavori di ricostruzione effettuati negli ultimi sette anni con l'impiego consistente di risorse pubbliche, al fine di verificare il corretto operato. Sono quindi molteplici le motivazioni che rendevano e rendono urgente la discussione in Aula di questo provvedimento, calendarizzato una prima volta a luglio, slittato a dopo la pausa estiva e

ma in una posizione che ne preclude la discussione, visto che stiamo esaminando un provvedimento corposo come quello riguardante le aree protette. Non solo, la speranza di poterlo discutere svanisce anche la prossima settimana

nella quale nelle settimane scorse è stata presentata una istanza per modificare gli impianti attraverso il cambiamento del combustibile

ma anche interpretando la legge in modo molto restrittivo e lacunoso, come purtroppo è successivamente emerso dall'esame degli atti. Ciò in particolare relativamente al fatto che è stata accuratamente evitata una nuova autorizzazione integrata ambientale, che invece, in questi casi, ad avviso di tutti, è assolutamente necessaria per valutare compiutamente gli effetti di questo cambiamento e, soprattutto, per le prescrizioni necessarie ad evitare effetti negativi sul piano dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni in atmosfera. Si è creata in questo Paese, che tra l'altro si trova all'interno di un parco, una situazione di elevato allarme sociale da parte dei cittadini, che rende assolutamente necessarie la sospensione dell'autorizzazione già data dalla commissione tecnica provinciale ambiente e la predisposizione di una nuova procedura

chiedendo una risposta cortesemente sollecita, vista la situazione di grande tensione sociale che da settimane vive la comunità dei cittadini a Monselice.